Signora Presidente, onorevoli senatori, ricordo ancora una volta che il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva in breve, il Piano d'azione per l'infanzia - è lo strumento di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. L'ultimo Piano d'azione adottato dall'Italia è quello del 2004 ed è quindi quanto mai avvertita l'esigenza di disporre di questo strumento, che costituisce il programma di lavoro, ratificato al più alto livello, frutto dell'esito del confronto tra le istituzioni centrali dello Stato, le Regioni, gli enti locali, le formazioni sociali e tutti gli altri attori impegnati nella promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi, per la realizzazione di interventi culturali, normativi ed amministrativi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, da realizzarsi a tutti i livelli di governo con la partecipazione attiva della società civile e in stretto raccordo con le istituzioni dell'Unione europea. Giunti ormai in dirittura d'arrivo, vorrei riassumere le tappe di questo percorso. Nell'autunno del 2007 l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, in seduta plenaria, ha approvato la prima bozza schematica - il telaio del piano da elaborare predisposta dal comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. All'interno dell'Osservatorio sono stati quindi individuati sette gruppi di lavoro su tematiche e contenuti specifici, ritenuti di interesse comune per le amministrazioni pubbliche, le formazioni sociali e i soggetti collettivi attivi nella promozione e nella difesa dei diritti dei bambini: il patto intergenerazionale e intragenerazionale; il il diritto alla partecipazione e ad un ambiente a misura di bambino; la povertà dei bambini e degli adolescenti; i minori verso una società interculturale; i minori rom, sinti e camminanti; il sistema delle tutele, delle garanzie e dei diritti; la rete dei servizi integrati. Una metodologia di lavoro collegiale ha quindi accompagnato tutte le fasi elaborative del Piano, il cui percorso di costruzione, coordinato dal comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale, è stato caratterizzato da una diffusa e articolata consultazione tra tutti i componenti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia che hanno partecipato ai gruppi e, per quanto possibile, con i soggetti collettivi che essi rappresentano e dalla concertazione nello sviluppo degli obiettivi strategici e nella armonizzazione delle politiche, dei servizi e degli interventi. Nel 2008 i gruppi di lavoro hanno terminato i propri lavori elaborando, per ogni ambito di intervento, una ricognizione sullo stato del dibattito e delle esperienze, un documento programmatico contenente obiettivi generali e specifici ed indirizzi progettuali per la realizzazione delle politiche a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Ricordo anche che non vi è stata soluzione di continuità nel lavoro dell'Osservatorio, perché esso era già stato insediato dal precedente Governo Prodi ed ha continuato ad operare nella continuità dei membri che erano stati a suo tempo insediati. Come concordato nella riunione plenaria dell'Osservatorio tenutasi nel febbraio 2009, si è quindi svolta, sempre all'interno dei gruppi, una fase di approfondimento e di individuazione delle azioni da realizzare, i cui risultati sono stati consegnati al comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

di approfondimenti sia da parte di membri del comitato sia da parte del Governo. Si è proceduto quindi, in particolare, alla verifica della coerenza delle azioni poste in capo alle amministrazioni centrali con gli indirizzi governativi, al fine di sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri, prevista dalla procedura per l'adozione del Piano, un testo il più possibile condiviso. Se dunque la necessità di questo confronto ha richiesto un tempo maggiore rispetto al previsto per la definizione del documento finale da sottoporre all'Osservatorio, la consultazione

consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale: è il "contenitore" di un sistema di intervento che dà continuità alle azioni di prevenzione, cura e recupero. Tra le azioni proposte in questo ambito vi sono quelle riguardanti il consolidamento del sistema dei servizi educativi per l'infanzia, il sostegno alla genitorialità alle famiglie con minori disabili, gli interventi sulle strutture di accoglienza per minori e la promozione dell'affidamento familiare, la prevenzione e la cura Ricordo che tutte queste tematiche, dopo la costituzione del 2001, sono da trattare di intesa tra le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, che hanno competenze in materia. In secondo luogo, occorre rafforzare la tutela dei diritti: è il settore di intervento centrato sulla protezione e sulla tutela prevalentemente giuridica. Fanno capo, tra le altre, a questa direttrice le indicazioni per la riforma del tribunale dei minorenni e dei procedimenti civili in materia di famiglia e minori, l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, le linee di indirizzo per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. In terzo luogo, va favorita la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale: è l'ambito di intervento che ha raccolto i contributi progettuali dei gruppi centrati sul protagonismo dei cittadini in crescita. Il tema della partecipazione è fortemente legato al tema del dialogo fra generazioni. I rapporti tra le generazioni, oggi, sono sicuramente influenzati dalla persistenza di un basso livello di natalità, dal continuo processo di invecchiamento della popolazione, dagli indubbi cambiamenti registrati nelle strutture e nei comportamenti familiari con la crescita di nuove e diverse tipologie di famiglie e da un persistente livello di alta disoccupazione giovanile. La promozione e la salvaguardia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza richiedono dunque un rapporto significativo con le generazioni adulte, a cui è chiesta un'assunzione diffusa di responsabilità, a cominciare - è evidente - dalle buone relazioni familiari, soprattutto con i genitori. Tra le azioni previste in questo ambito, oltre a quelle destinate a costruire e sostenere i rapporti tra le generazioni, stanno quelle finalizzate al miglioramento della qualità dell'evento nascita e a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Registro con soddisfazione che secondo il recentissimo rapporto di «Save the children» l'Italia è il primo Paese al mondo per basso indice di mortalità infantile, il Paese cioè in cui vi sono meno morti nel momento del parto. promuovere l'interculturalità: è la direttrice in cui sono confluite le proposte riguardanti i minori stranieri ed i minori rom, in particolare per quanto riguarda la prevenzione della dispersione scolastica, il sostegno e l'accompagnamento educativo, ma anche il sostegno alle seconde generazioni. Più di un quinto dei 3.900.000 stranieri residenti in Italia è minorenne, e ciò è indice del carattere sempre più stabile e radicato che l'immigrazione sta assumendo in Italia. Per società interculturale si intende una comunità che non rinuncia alla sua identità culturale e valoriale, ma favorisce con intelligenza i processi d'integrazione degli individui e dei gruppi di immigrati, definendo un progetto teso a costruire nuove relazioni e interconnessioni. Le giovani generazioni sono chiamate a costruire una convivenza plurietnica, avendo come riferimento valori fondamentali su cui l'impegno sociale e istituzionale e l'educazione non possono non possono non convergere: il rispetto della democrazia, il rispetto della legalità, il rispetto della persona, il rispetto della famiglia, il rispetto delle diversità, il rispetto dei sentimenti e, naturalmente, l'adesione ai nostri principi costituzionali. Per ognuna di queste direttrici si sono individuate le problematiche principali e gli obiettivi generali, che sono stati arricchiti dai contributi derivanti dalle conclusioni dei gruppi di lavoro tematici organizzati in occasione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, svoltasi a Napoli dal 18 al 20 novembre 2009. Contiamo, a questo punto, di presentare al più presto (*ad horas* direi) all'Osservatorio la stesura definitiva del Piano. Tutto ciò premesso, ed entrando maggiormente nel merito, va detto che il Piano non è un mero adempimento rituale, ma si pone l'ambizioso obiettivo di operare come uno strumento innovativo. Elementi di continuità e di discontinuità con le impostazioni dei Piani precedenti lo caratterizzano non solo come un nuovo Piano d'azione, ma come un Piano con caratteristiche nuove. La continuità riguarda innanzitutto il permanere della necessità di dare unitarietà e coerenza alle scelte e alle politiche del Governo per l'infanzia e l'adolescenza e, di conseguenza, alle politiche ed ai servizi, evitando scollamenti e frammentazioni tra gli interventi. secondo luogo, si vuole continuare e incrementare la costruzione di una cultura della cooperazione tra istituzioni pubbliche e realtà del privato sociale, in linea con la riforma costituzionale del 2001, Vanno emergendo lentamente prospettive positive e creative che stanno dando vita in punta di piedi ad un nuovo diritto minorile, che nasce dai territori e si propone in termini nuovi. La discontinuità riguarda, invece, principalmente due dimensioni. Rispetto all'approccio, il presente Piano non affronta tutto il complesso delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, ma ha identificato alcune dimensioni prioritarie che rappresentano le direttrici di intervento sulle quali ha sviluppato proposte ed azioni coordinate. Le priorità individuate hanno inteso sottolineare l'attenzione ad alcuni aspetti ritenuti importanti, ma non hanno voluto affatto proporre delle tematiche settoriali, tendendo piuttosto a pervenire alla globalità dell'analisi e alla trasversalità delle azioni partendo dalle priorità indicate. dalle priorità indicate. Rispetto al metodo, la peculiarità è rappresentata dalla scelta di adottare un processo partecipato non solo nella fase della costruzione del Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, ma anche della sua attuazione attraverso la programmazione di un percorso di accompagnamento e di monitoraggio permanenti, con l'obiettivo di favorire la sua corretta applicazione e valutazione. Un percorso di affiancamento che impegnerà tutte le componenti del settore pubblico e della società civile. Va ricordato che il Libro bianco presentato dal ministro Sacconi sul futuro del modello sociale, approvato dal Consiglio dei ministri il 6 maggio 2009, orienta la riforma del *welfare* italiano secondo un modello sociale volto a promuovere l'autosufficienza di ciascuna persona, sia come individuo sia come parte delle formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia. Il primo valore guida in questa sfida è proprio quello costituzionale della centralità della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali: la famiglia, quale luogo delle relazioni affettive; il lavoro, quale espressione di un progetto di vita; la comunità e il territorio, quali ambiti di relazioni solidali. Da questo valore discende un *welfare* delle opportunità e delle responsabilità che si rivolge alla persona nella sua integralità, destinato progressivamente a sostituire il modello attuale di tipo prevalentemente risarcitorio. Un *welfare* che interviene in anticipo, con un'offerta personalizzata e differenziata rispetto al formarsi del bisogno e che sa stimolare comportamenti e stili di vita responsabili e, per questo, utili a sé e agli altri. Un modello sociale così definito si realizza non solo attraverso le funzioni pubbliche, ma anche riconoscendo, in sussidiarietà, il valore della famiglia, della impresa profittevole e non, come di tutti i corpi intermedi che concorrono a fare comunità. L'approvazione dello schema di Piano d'azione da parte del Governo costituirà l'avvio della fase di attuazione, che sarà caratterizzata dalla coprogettazione, dalla cogestione e corresponsabilità e dal controllo partecipato. La coprogettazione, consisterà in una progettazione operativa partecipata, condivisa, trasparente e scandita da momenti pensati, dedicati, specifici, espliciti e verificabili nei quali sono coinvolti i diversi soggetti interessati. La cogestione/corresponsabilità, nella diversità e nel rispetto di ruoli e funzioni, riguarderà le varie azioni, sia a livello centrale che territoriale. Il controllo partecipato consisterà nell'accompagnamento, nel monitoraggio e nella valutazione degli esiti delle azioni proposte dal Piano d'azione, che vedrà coinvolti lo stesso Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale, oltre che la collegialità dei soggetti impegnati nella realizzazione del Piano. Consentitemi, in conclusione, di ricordare che la prossima approvazione dello schema di Piano da parte dell'Osservatorio nazionale l'infanzia e l'adolescenza prelude *ex lege* ad un'ulteriore, laboriosa fase di confronto ed elaborazione. Il Piano dovrà essere infatti portato all'esame preliminare dei Consiglio dei ministri, dopodiché approderà, per il prescritto parere, alla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza e poi alla Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali. Dunque, la procedura prevede che il dibattito e la possibilità di arricchire lo schema di Piano siano i più ampi possibili, con l'apporto non solo delle amministrazioni centrali, ma anche del Parlamento e del sistema delle autonomie. Solo dopo questi passaggi il Piano tornerà in Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione e sarà poi adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Un cenno va fatto, infine, alle modalità di finanziamento degli interventi previsti nel Piano: in alcuni casi si tratta di azioni e interventi a costo zero o finanziabili nei limiti di stanziamenti già previsti. Dove si renderà necessaria la presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi, occorrerà valutarne gli oneri e reperire la copertura finanziaria. In generale, agli impegni contenuti nel Piano che, ricordo, è Piano non solo del Governo centrale, ma di tutti i livelli di governo - è da riconoscere carattere programmatico e non immediatamente operativo. Ciononostante, dichiaro qui la mia disponibilità a destinare ad alcune delle azioni previste, e nel rispetto del criterio della condivisione con le Regioni ed il sistema delle autonomie locali, anche parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia.

signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, ringrazio il Governo per l'esposizione del III Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e per la scelta di indirizzi e di priorità che vedo sviluppata in questo Piano, con azioni, come ha appena ricordato il Sottosegretario, che dovranno essere giustamente concertate con le Regioni e gli enti locali per la cogestione e la corresponsabilità. Apprezzo molto il rafforzamento della rete di servizi e di operatori per un vera presa in carico globale del bambino e della sua famiglia. un ampio spazio dedicato alla centralità della famiglia come pilastro della nostra società. Il Sottosegretario ha menzionato lo spazio dedicato alla scolarizzazione ed al rafforzamento della tutela dei diritti dell'infanzia. I 10 milioni di bambini e ragazzi italiani sono una risorsa unica per il nostro Paese, e voglio qui riprendere una dichiarazione del 1997 del segretario dell'ONU Kofi Annan, quale affermava che il mondo di domani sarà influenzato dalla scienza e dalla tecnica, ma sta già prendendo forma nei corpi e nelle menti dei nostri figli. Importante in questo Piano è l'intervento di rafforzamento dei servizi di accompagnamento della genitorialità, promuovendo interventi educativi domiciliari, che poi penso verranno esposti in modo più preciso dinanzi alla Commissione bicamerale per l'infanzia. Ho apprezzato molto la doverosa attenzione che, per i cambiamenti socio-culturali, si pone per la costruzione di un patto intergenerazionale, con la condivisione dell'educazione tra la famiglia (purtroppo non sempre consapevole della sua responsabilità educativa), la scuola e la società. A questo proposito in Commissione infanzia stiamo valutando proprio gli effetti negativi di determinate azioni azioni della società, soprattutto, ad esempio, della Rete e della sua pericolosità come mezzo di informazione e talora come metodo di adescamento dei minori.

Il nostro Paese, come tantissimi altri nel mondo, ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ma la sua azione non è conseguente: troppe sono le mancanze ed avremmo bisogno di una svolta nella cultura dell'infanzia, nelle leggi, negli investimenti. La vita dei bambini, i loro bisogni, i loro diritti, il loro presente ed il loro futuro devono diventare priorità del Paese. Le famiglie devono essere sostenute nella crescita dei figli. È necessario un progetto lungimirante, un coordinamento delle azioni pubbliche e private, una valorizzazione delle competenze dei bambini e degli adolescenti, delle famiglie, delle associazioni e delle professioni. Continuiamo a spendere meno della metà della media europea per i bambini e gli adolescenti e, nonostante negli ultimi anni si siano aggravate le condizioni di vita di tanti bambini, in particolare al Sud, il Governo ha tagliato tante risorse per l'infanzia e l'adolescenza. Le conseguenze sono per l'Italia il persistere di uno dei più bassi tassi demografici al mondo, di un tasso di povertà minorile tra i più alti d'Europa e di un tasso di dispersione scolastica tra i più alti: l'ultimo provvedimento del Governo ha abbassato l'obbligo scolastico a 15 anni, mentre in Europa si va verso i 18 anni. Esiste una grande disparità nelle risorse e nei servizi tra Nord e Sud, e la riforma federalista dello Stato, senza una legge quadro dell'infanzia e dell'adolescenza che indichi i livelli essenziali e le priorità, può aggravare le diseguaglianze sociali e territoriali.

Ci sono Regioni, come la Toscana, l'Emilia-Romagna, l'Umbria e tante altre, tra cui alcune del Nord, che hanno superato di gran lunga il 33 per cento, ma il Governo ha tagliato tutti i fondi. nidi sono insufficienti non solo per mancanza di investimenti, ma perché si sottovaluta la loro importanza per lo sviluppo della personalità dei bambini. Non ci sono servizi adeguati per contrastare nuove e vecchie forme di disagio - dall'obesità (la più alta in Europa), all'anoressia e alla bulimia - e per accompagnare le varie fasi della vita, a partire dall'adolescenza. C'è oggi più disattenzione, che arriva fino all'indifferenza e anche al fastidio, nei confronti dei bambini disabili e dei migranti. Non si sviluppano servizi adeguati per rendere più semplice l'adozione e l'affido; manca ancora la banca dati. E non ci si attrezza in modo convincente, così come richiesto dall'Organizzazione mondiale della sanità

I bambini italiani sono oggetto del doppio degli *spot* rispetto agli altri Paesi europei. È poi venuta meno l'attenzione alla cooperazione internazionale rivolta ai bambini. La crisi ha colpito in particolare le famiglie con figli, ed è dai loro diritti che bisogna ripartire, anche con politiche fiscali adeguate. Si continuano a scindere i temi dello sviluppo economico da quelli della cura delle persone:

questo ci chiedono i cittadini; questo è necessario per il presente e il futuro dell'Italia. Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, condividiamo che il primo valore guida che deve dirigere l'azione della politica nella tutela dei minori è quello costituzionale, che vede la centralità della persona, in sé e nelle e nelle sue proiezioni relazionali; la famiglia, quale luogo delle relazioni affettive ed educative; il lavoro, quale espressione di un progetto di vita; la comunità ed il territorio, quali ambiti di relazioni solidali. Il Piano nazionale degli interventi per la tutela dei minori è lo strumento di attuazione della Convenzione affinché si realizzino interventi culturali, normativi ed amministrativi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. È positivo che tale Piano coinvolgerà lo Stato, le Regioni, gli enti locali, la scuola e tutti gli attori impegnati nella promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi. Al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave sottosviluppo, dove essi sono costretti a combattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili, vengono sottoposti ad abusi sessuali o a violenze punitive, cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento: i diritti dei bambini sono violati anche in quei Paesi che hanno raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati. Nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono spesso connessi a profondi problemi culturali e a gravi carenze economiche nell'ambito familiare oltre che all'ondata dei flussi migratori clandestini. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di estrema fragilità causata dallo stato di illegalità in cui si trovano, diventano facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali: dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità. Per queste ragioni la Lega Nord ritiene di fondamentale importanza perseguire una linea politico-programmatica incentrata da un lato nel contrasto all'immigrazione clandestina e dall'altro lato nel nel potenziamento di quelle attività volte a sviluppare un modello di integrazione basato sul rispetto dei medesimi doveri e sul godimento degli stessi diritti. La promozione dell'interculturalità non può non passare dalla valorizzazione della nostra cultura e delle nostre tradizioni. La consapevolezza della ricchezza dei valori di cui siamo portatori e che tali valori non possono e non devono essere negoziabili, ci permetterà di sostenere azioni forti e positive a sostegno dei minori portatori di culture diverse e di tutti i minori in difficoltà. Dunque, la strada da seguire è quella della presa di coscienza che nel nostro Paese c'è una cultura valoriale di riferimento che non può accettare continue deroghe. In Italia è esposto a rischio di povertà il 24 per cento dei minori, quasi uno su quattro. Tale percentuale raggiunge il 40 per cento nel caso di minori che vivono in famiglie monoparentali. I minori più a rischio sembrano essere quelli che vivono in famiglie con entrambi i coniugi lavoratori ma i cui bassi livelli di reddito non riescono ad essere una garanzia Per quanto concerne i bambini e gli adolescenti particolarmente vulnerabili ai numerosi fenomeni di sfruttamento e abuso, la Lega Nord chiede l'impegno ad un monitoraggio sempre più articolato delle criticità, al fine di individuare in modo puntualmente mirato le politiche di contrasto più efficaci. Dunque, i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia debbono essere: la conoscenza del problema in tutte le sue sfumature, il coinvolgimento attivo della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel territorio, la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola sono certamente i primi ambiti dove i bambini possono conoscere i valori della partecipazione, della tutela, della condivisione e del senso di appartenenza. Siamo convinti come Lega Nord che l'autonomia impositiva regionale e locale disegnata dalla nuova legge delega sul federalismo fiscale è diretta a superare la logica dei trasferimenti vincolati, ad alto tasso di burocrazia e a basso tasso d'incidenza sullo sviluppo reale, e ad aprire così una nuova stagione anche anche per la tutela della famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale sarà guidata secondo i princìpi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Si tratta di princìpi altamente innovativi, che connotano questa riforma del federalismo fiscale nella direzione di un maggiore riconoscimento fiscale dei carichi familiari Concludo dicendo che apprezziamo il contenuto del Piano qui anticipato dal sottosegretario, senatore Giovanardi e con una battuta: una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come insegna Aristotele, una buona politica non afferma princìpi, ma propone risposte fattibili a problemi concreti.

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia ha compiuto vent'anni. Tuttavia, nonostante questo accordo abbia ormai ampiamente raggiunto la maggiore età, dobbiamo constatare purtroppo che molte disposizioni in essa contenute non hanno ancora trovato nel nostro Paese una piena applicazione. Innanzitutto, non è stata messa a punto una riforma del sistema di giustizia minorile per la quale si dovrebbero prevedere: competenze esclusive in capo ad un unico organo specializzato; una riforma della normativa relativa alla difesa d'ufficio, in modo tale da consentire un'effettiva applicazione della legge 149 del 2001 nella parte che prevede la difesa tecnica del minore nelle procedure di adottabilità e *de potestate*; una riforma dell'ordinamento penitenziario minorile. Per quanto riguarda le politiche sociali, è da segnalare la mancata definizione in maniera concorrente tra Stato e Regioni dei livelli essenziali di prestazioni sociali (i cosiddetti LIVEAS) che crea di fatto un grave vuoto legislativo. Infatti, in base al Titolo V della Costituzione, la competenza in materia di politiche sociali è affidata alle Regioni: la mancata individuazione di standard minimi nazionali potrebbe comportare la possibilità che tutto venga affidato a decisioni totalmente discrezionali da parte delle singole Regioni sull'unica base delle risorse regionali disponibili, con il rischio concreto di creare pesanti sperequazioni nei servizi erogati. Tra l'altro, il fatto che il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 285 del 1997, sia confluito al 70 nel Fondo nazionale per le politiche sociali, stabilito dalla legge n. 328 del 2000, (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), crea un'ulteriore disparità tra le 15 città cosiddette riservatarie, che continueranno ad usufruire del restante 30 per cento del Fondo triennale per l'infanzia e l'adolescenza, ed il resto del territorio nazionale. Poiché lo Stato centrale ha comunque la responsabilità di garantire l'uniforme godimento dei diritti da parte di tutti gli individui sul territorio nazionale, sarebbe fondamentale la stipula di un atto d'intesa tra Stato, Regioni e autonomie locali sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, come richiesto anche da numerose associazioni del settore, sarebbe necessario introdurre un sistema di monitoraggio per analizzare annualmente l'entità delle risorse italiane destinate all'infanzia e all'adolescenza, tenendo conto delle risorse stanziate dai diversi Ministeri competenti, dalle Regioni e dagli enti locali. Anche il Piano nazionale dell'infanzia rientra tra i mancati adempimenti dell'Italia. In base alla legge n. 451 del 1997, il Piano dovrebbe essere predisposto ogni due anni dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, sentita la relativa Commissione bicamerale, ed approvato dal Consiglio dei ministri. Finora invece l'unico Piano nazionale approvato continua ad essere quello relativo al biennio 2002-2004. Nel 2007 l'Osservatorio nazionale l'organo che è incaricato di predisporre il Piano nazionale fornendo indicazioni rispetto ai contenuti ed alle modalità con cui dovrebbe essere elaborato tale documento, era stato ricostituito e riorganizzato. I lavori dell'Osservatorio, che avrebbero dovuto portare alla predisposizione del Piano entro il mese erano stati interrotti dalla fine della XV legislatura e ripresi di fatto solo il 26 febbraio 2009, definendo come termine ultimo il successivo mese di giugno 2009 per l'approvazione definitiva del Piano. Nella bozza di piano originaria erano individuate precise direttrici d'azione ispirate ai principi della Convenzione ONU: favorire la partecipazione dei minori per la costruzione di un patto intergenerazionale; promuovere l'interculturalità; consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale; rafforzare la tutela dei diritti. Dopo quasi due anni di lavoro, tuttavia, in maniera incomprensibile considerato anche il ritardo già accumulato, il Governo annunciava che l'approccio culturale del Piano proposto dall'Osservatorio non era condivisibile e decideva, di fatto esautorando l'Osservatorio stesso, di predisporre una propria proposta basata, sulla maternità, sulla famiglia e sulle relazioni familiari. Sembrerebbe che il Governo, per motivi puramente ideologici e non tenendo conto dell'evoluzione del concetto di famiglia, stia di fatto confondendo le politiche per la famiglia con quelle per i minori. Si rileva

il Piano alla competente Commissione bicamerale e assicuri adeguati finanziamenti per la sua implementazione, oltre ad un adeguato coordinamento con il livello regionale delle azioni ed interventi previsti. Nel ringraziarla, signor

anche - altre colleghe l'hanno detto - che l'ultimo Piano approvato dal Governo risale agli anni 2002-2004. Il Governo si è già impegnato, anche in occasione della Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza tenutasi a Napoli lo scorso novembre 2009, a proseguire

Serve un progetto educativo che coinvolga scuole, associazioni, genitori; in sostanza la famiglia. La famiglia deve essere la prima fonte di educazione alla vita e, naturalmente, il ruolo educativo della scuola è

il Governo ritiene di aver esercitato il massimo rispetto per il Senato. Ne prendiamo atto. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.